dipende da questioni socio‑economiche. I fattori principali che hanno una correlazione positiva con la crescita dell'obesità

In particolare, con la mozione in esame vogliamo sensibilizzare i colleghi e l'Assemblea intera sulle politiche di comunicazione che si possono fare per ridurre o quanto meno per tentare di ridurre in prospettiva il fenomeno.

ormai rilevante sulla borsa della spesa l'iniziativa dei bambini e degli adolescenti, molto più elevata di quella dei genitori. quindi opportuno agire in tal senso. Lo stesso tipo di azione viene fatta negli Stati Uniti. Oltretutto, noi viviamo un po' il mito della dieta mediterranea. Non passa settimana in cui non esca un articolo su qualche giornale che parla bene di questa dieta; messa così, potremmo essere d'accordo tutti, però, dieta mediterranea non vuol dire mangiare mezzo chilo di pasta. Lo dico da

Sono cose molto semplici, che però servono per istruire i nostri ragazzi ad un tipo di alimentazione più salutare e, in prospettiva, più sana per tutto il Paese.

merendine o altro, che può fare male e molto ai ragazzi, perché se si diventa in sovrappeso o, peggio ancora, obesi in età infantile è poi molto più difficile ritornare in linea quando si è adulti.

Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, sono già state illustrate alcune delle motivazioni che hanno indotto alcuni Gruppi al Senato a presentare una mozione sull'obesità infantile. La necessità di dibattere sull'obesità infantile è riconosciuta ormai - come ricordava il collega Garavaglia - dai maggiori Paesi europei, il cui Governo ha approntato un piano d'azione veramente notevole. Per noi diventa importante stabilire quali possono essere le linee d'azione per un piano efficace di prevenzione e di cura dell'obesità infantile.

È possibile intervenire su di esse? Se guardiamo i dati e le previsioni, anche in relazione al contesto europeo, ci rendiamo conto degli elementi preoccupanti. L'Italia è ai primi posti in Europa per il numero di bambini in sovrappeso, e i dati sono destinati a peggiorare, in quanto in Europa il sovrappeso in età scolare cresce al ritmo di circa 400.000 casi all'anno.

Riportando questi valori a tutta la popolazione di bambini di età sei-undici anni si giunge ad una stima di più di un milione di bambini sovrappeso od obesi in Italia. Analizziamo le conseguenze dell'obesità sulla salute psicofisica dei bambini. alcuni aspetti della realtà della salute: dal 30 al 60 per cento dei bambini obesi mantengono l'eccesso ponderale in età adulta e presentano più frequentemente del previsto alterazioni metaboliche e complicanze rispetto all'obesità che si manifesta in età adulta. Anche per quanto concerne le conseguenze sulla salute psichica vediamo che, nel contesto culturale dei Paesi occidentali, il bambino obeso può sviluppare un disagio psicologico che può contribuire all'instaurarsi di un disturbo del comportamento alimentare. È stato stimato che in età pediatrica sono presenti per il 3,5 per cento; inoltre, una recentissima indagine mette in evidenza la stretta relazione che intercorre tra bassa autostima e eccesso di peso nei bambini obesi.

al rapporto tra pubblicità nell'offerta alimentare rivolta ai bambini e obesità infantile. Da una ricerca americana emerge che, per quanto riguarda i danni della pubblicità sulla salute dei minori, in base agli studi condotti, il divieto di *spot* di *fast food* nei programmi per bambini e ragazzi ridurrebbe del 18 per cento il tasso di obesità dei bambini e del 14 per cento degli adolescenti statunitensi. Non a caso gli *spot* pubblicitari nei programmi per bambini sono vietati anche in molti Paesi europei: in particolare in Svezia, Norvegia e Finlandia, ma non solo; sono regolamentati anche in Inghilterra, Francia e Germania.

di insistere ormai da un decennio sul legame strettissimo tra pubblicità e obesità infantile e di aver indirizzato richieste e raccomandazioni

sull'influenza della televisione sui comportamenti degli adolescenti dimostra che la visione della TV incide fortemente sull'abitudine alimentare dei bambini: più televisione si guarda, più si mangiano solo le cose che piacciono, più aumenta nettamente il consumo di merendine confezionate, mentre cala già basso consumo di verdura e aumenta il consumo di dolci e salumi. Vorrei citarvi i seguenti questi dati: un bambino italiano che guarda una media di tre ore di televisione al giorno subisce circa 32.850 pubblicità di alimenti nell'arco di un anno; in sostanza una ogni cinque minuti. In complesso, sono state sottoposte ad analisi 24 reti televisive in 11 Paesi europei. Dallo studio è emerso che la situazione italiana appare peggiore della media europea. Le differenze numeriche tra i Paesi considerati sono significative: la Svezia, ad esempio, trasmette solo un quindicesimo degli *spot* trasmessi in Polonia e circa un decimo di quelli trasmessi in Italia. Se poi si entra nei contenuti dei messaggi trasmessi, si vede che in Italia gli *spot* che pubblicizzano alimenti ricchi di zuccheri, grassi e sali, quindi ipercalorici, interessano il 36 per cento della pubblicità e ovviamente nessuno *spot* ammonisce circa il corretto consumo di tali cibi. Al contrario, l'idea di usare la pubblicità per insegnare a mangiare bene è una pratica utilizzata in Paesi come Spagna, Gran Bretagna, Polonia e Portogallo. Alla Alla luce di queste considerazioni, si ritiene di fondamentale importanza ribadire la necessità di un sistema di limitazioni normative per la pubblicità commerciale, mirate agli obiettivi di tutela dei minori, che li proteggano dagli effetti dannosi e nello stesso tempo valorizzino la produzione di qualità.

ad affrontare un prima tema che è la tutela dei bambini nella pubblicità. La seconda grande questione riguarda lo sport nella scuola, l'alimentazione e la scuola. Anche in caso abbiamo una grande necessità di prevedere un'azione lungimirante e decisa per quanto riguarda il mondo della scuola; abbiamo la necessità di farlo perché la scuola diventa un punto di riferimento importantissimo. Dobbiamo prevedere misure di prevenzione dell'obesità infantile: insegnanti, medici scolastici, personale della ristorazione scolastica, personale specializzato nella cura e negli studi dell'età prescolare debbono fare corsi di formazione. Risulta, quindi, necessario integrare l'alimentazione e la nutrizione nella maniera più concreta possibile nel programma scolastico;

formare gli insegnanti perché possano aiutare più efficacemente gli allievi alla lettura critica della pubblicità; dare forza vincolante alle raccomandazioni volte a organizzare la ristorazione scolastica (aspetti nutrizionali, educativi, reperimento dei pasti) ed estenderle a tutte le forme di ristorazione collettiva frequentate dai giovani; mettere a disposizione dell'acqua gratuitamente e offrire l'opportunità di consumare frutta fresca in tutti i luoghi pubblici frequentati dai bambini, iniziando, per esempio,

C'è tutta una parte che riguarda la scuola e l'alimentazione che può essere approfondita e che noi e che noi descriviamo anche nel dettaglio nella mozione e a cui rimando. L'altra grande questione riguarda la salute della madre e dei bambini dalla nascita fino all'età di tre anni.

avere un *target* che sono le donne in gravidanza e privilegiare tutti gli attori che sono coinvolti in questa azione di prevenzione. Un'attenzione particolare va rivolta alle famiglie di un ambito socio-economico sfavorevole; occorre sensibilizzare le donne in età fertile sui benefici che possono essere tratti

ma certamente risulta opportuno sviluppare una politica alimentare attraverso un'articolazione istituzionale che permetta di migliorare le politiche agricole, le politiche economiche, dell'educazione, di sanità, di ricerca; sviluppare il consumo di frutta e di verdura facendo leva sulle loro qualità organolettiche e gustative, la loro reperibilità, la loro accessibilità e attrattiva, sviluppando le filiere di produzione con l'obiettivo di eliminare

molteplici aspetti che la causano; pertanto la risposta non può che prevedere molteplici azioni. Per questo è indispensabile, come hanno fatto grandi Paesi, un piano di azione complessivo che sia in grado di attivare tutti gli attori a partire dal mondo economico, dal mondo delle istituzioni, dal mondo scolastico fino ai diversi Ministeri. Solo con un piano d'azione che che sia in grado di intervenire in tutti i settori, attraverso una gerarchia di intervento e con una articolazione anche nel tempo, possiamo affrontare efficacemente questo gravissimo problema.

D'altro canto, vi sono Paesi sviluppati che nei confronti dei bambini si comportano allo stesso modo, cioè non educano i bambini all'alimentazione e, anzi, l'alimentazione diventa un modo di sfuggire

Gruppo dell'Italia dei Valori siamo allarmati dai dati che tutti i giorni vengono diffusi dai vari organi competenti in materia di obesità infantile e che sono stati illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto; preoccupanti sono infatti le conseguenze di tale obesità sulla salute non solo nel corso dell'infanzia, ma anche nell'età adulta. Non sono un medico, ma è noto che tali conseguenze, se sottovalutate, rischiano di essere davvero disastrose. Le prime manifestazioni cliniche di obesità infantile si presentano a carico dell'apparato respiratorio, con affaticamenti e apnea notturna, e dell'apparato locomotore con dolori articolari, mobilità ridotta e piedi piatti. Assai grave è inoltre il rischio che il bambino obeso possa sviluppare un disagio psicologico, che può contribuire a sua volta all'instaurarsi di un disturbo del comportamento alimentare, e gli eventuali disagi psicologici sviluppati in età adolescenziale possono acuirsi e peggiorare nell'età adulta. Da adulto, il soggetto obeso fin da bambino, rispetto a chi è diventato obeso successivamente, risulta maggiormente esposto ad una serie di patologie, da quelle a carico dell'apparato cardiocircolatorio a quelle e dell'apparato muscolo-scheletrico a quelle di tipo metabolico, come il diabete mellito e l'ipercolesterolemia. È indubbio che la diffusione dell'obesità infantile, pur costituendo un problema sanitario a tutti gli effetti, affonda ancora le proprie radici in abitudini sociali ed approcci culturali che non tengono in alcun conto l'educazione alimentare. Dal punto di vista socio-culturale è facilmente rilevabile come scelte alimentari spesso inadeguate alle effettive esigenze dell'infanzia, inclini ad assecondare gusti e preferenze dei bambini piuttosto che ad orientarne le scelte verso alimenti sani e nutrienti, siano tra le maggiori cause della diffusione dell'obesità e del sovrappeso dei bambini; a ciò si deve purtroppo aggiungere l'impatto molto negativo di taluni messaggi pubblicitari specialmente attraverso il mezzo televisivo. La pubblicità di alimenti non sani effettuata in determinate fasce orarie e, in modo particolare, nel corso di programmi televisivi rivolti ad un pubblico di bambini o adolescenti costituisce, secondo recenti studi sia europei che americani, un potente veicolo di diffusione di quelle abitudini alimentari errate che costituiscono il presupposto per il diffondersi dell'obesità.

Nel corso di tale audizione i rappresentanti della SIP (professor Luigi Cataldi e dottor Maurizio Tucci) hanno sottolineato come la visione della TV incida fortemente sulle abitudini alimentari dei bambini e dei minori in generale.

Spesso, come sottolineano i rappresentanti della SIP, gli alimenti pubblicizzati sono di aspetto appetitoso e gradevole ma probabilmente non ottimali per le diete dei ragazzi. Quasi sempre infatti si tratta di dolciumi o *snack* dolci o salati, alimenti ricchi di sale, grassi e zuccheri; un ruolo fondamentale e imprescindibile nel contrasto alla diffusione di errate abitudini alimentari spetta anzitutto ai genitori, cui va fornita un'adeguata informazione sui rischi che una errata alimentazione possono provocare al proprio figlio; è altresì fondamentale il ruolo dell'istituzione scolastica nella diffusione dell'educazione alimentare; l'obesità è un problema complesso a mettere a sistema un piano nazionale di azione per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile che coinvolga l'insieme degli attori sociali e che privilegi un approccio di promozione della salute e di stili di vita sani a porre in essere una concreta campagna di informazione riguardo l'alimentazione e la nutrizione, l'attività fisica, la lotta contro la sedentarietà,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, i numeri, le percentuali, le statistiche sul grave problema dell'obesità infantile nel nostro Paese sono stati ampiamente riportati riportati nelle mozioni. Non ci consola il dato che nei Paesi anglosassoni le percentuali sono più alte, che ben oltre il 50 per cento della popolazione complessiva americana risulta essere in sovrappeso. Anzi, ci preoccupa doppiamente, perché conferma un *trend* generalizzato nel mondo occidentale, che già oggi parla di un miliardo di persone in sovrappeso; doppiamente inquietante, quando questo dato coincide con un identico numero: un miliardo di persone che, al contrario, non hanno sufficiente cibo. Stiamo parlando di salute, certo, ma anche di un alto tasso di disumanizzazione in crescita, di una profonda ingiustizia globale, di uno squilibrio che se non incrocerà tanti risvegli di coscienze e di consapevolezze, tante sensibilità che si attivano è un *trend* destinato solo a crescere, ad allargare la forbice e le distanze tra due mondi, quello dove si «muore per mancanza» e quello dove si «muore per eccesso». E qui, nel secondo, nel nostro, proprio l'obesità e il sovrappeso derivanti da stili di vita non equilibrati sembrano essere le cause principali delle cosiddette patologie *killer*, che si stanno diffondendo in maniera sempre più massiccia. È stato ormai ampiamente dimostrato che, insieme ad una insufficiente attività fisica, è proprio un regime alimentare sbagliato la causa di molte patologie predisponenti al diabete, alle malattie vascolari, al cancro. Ne è causa principale una alimentazione in eccesso: troppa alimentazione, troppo carica di grassi e zuccheri, troppo povera di frutta e verdura. La gravità della situazione è talmente evidente che organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità la stessa Unione europea si stanno impegnando nella ricerca di indirizzi capaci di affrontare il problema di una nuova cultura alimentare. Per questo, partirà nei prossimi mesi il programma «frutta nelle scuole» anche nel nostro Paese, promosso dall'Unione europea insieme ai Ministeri delle politiche agricole e della sanità, finalizzato all'incremento di frutta nella dieta degli studenti della fascia primaria. In questi ultimi anni sono state analizzate le patologie insieme alle diverse diete alimentari del mondo, e anche da qui è emerso in modo inconfutabile che vi è correlazione stretta tra stile alimentare e salute ed è emerso come la dieta mediterranea risulti essere il modello più efficace in termini di benessere e prevenzione delle patologie croniche. Del resto, proprio quest'Assemblea, un anno fa, ha sostenuto il valore della dieta mediterranea. risulta anche che dagli anni Cinquanta ad oggi vi è stato, in tutta l'area del Mediterraneo, Italia compresa, un graduale abbandono di questa dieta a favore di stili alimentari meno salutari, con un parallelo aumento dell'obesità. situazione grave e lo è un po' di più da noi: nell'Italia delle eccellenze, delle DOP di frutta e verdura, non è solo grave, ma diventa un paradosso. Nel Paese delle più numerose varietà e delle qualità più alte di ortofrutta cala il consumo di frutta e verdura nelle diete dei bambini e dei ragazzi, i nostri futuri adulti. Nel Paese dove la mancata prevenzione alimentare registra costi sanitari in aumento - nell'ordine delle decine di milioni di euro, se vogliamo addirittura monetizzare il danno nello stesso Paese, nello stesso tempo e sugli stessi territori dell'emergenza sanitaria, per contro, il settore dell'ortofrutta vive una crisi fortissima con cali di vendite di prezzi ai produttori che raggiungono picchi del meno 20 per cento nel 2009 e diverse aziende stanno chiudendo. Credo sia molto difficile intervenire sui cambiamenti degli stili di vita, soprattutto quando ci si deve misurare con un bombardamento mediatico delle proporzione ben indicate nella mozione di cui è prima firmataria la senatrice Serafini. Certamente non bastano decreti e delibere, ma credo che non ci si possa neppure rassegnare all'insensatezza, alla stupidità dannosa che fa buttare le pesche nettarine in discarica, fa aumentare i fritti nei sacchetti delle merende a scuola, poi fa correre le madri dai medici e riempie i reparti pediatrici. Tutto questo mentre le aziende di ortofrutta non reggono. Di fronte a questa situazione deve esserci una saggezza più alta che deve partire proprio dalla politica, perché questo è il suo compito; una saggezza che ricerca il bene della salute e dell'economia nello stesso tempo e non lascia che si scivoli verso il danno di tutti solo per il *business* di pochi. pochi. Una saggezza ancora più utile - credo - in tempo di crisi. Allora se una presa di coscienza profonda c'è, sono d'accordo che occorre un piano straordinario per la prevenzione e la cura di lunga prospettiva. Ci sono azioni dentro questa scelta che si possono attivare da subito. Il progetto frutta nelle scuole è importante ma è sperimentazione: da evento episodico deve diventare prassi consolidata, modo di essere. Non è tutto da inventare: si era già avviato nella scorsa legislatura, promossa dall'allora Ministeri delle salute e della pubblica istruzione, un progetto «frutta *snack*» nelle scuole, che ha coinvolto in tre città

realizzato in modo strutturale, costante e continuo. Andrebbe ad incidere sulla salute di centinaia di migliaia di ragazzi, provocherebbe un cambiamento di stile alimentare; inciderebbe sullo stato di salute di centinaia di aziende di ortofrutta. Occorre un progetto, un fondo destinato alle scuole in modo che, insieme alle merende naturali, si vadano ad attivare iniziative di sensibilizzazione e, dico ancora, di iniziative di animazione, perché il consumare frutta non sia solo un'imposizione salutistica, non sia un metter lì la frutta. Deve essere una scelta accattivante; deve incrociare le reazioni dei ragazzi e il mangiare frutta, come dicono gli adolescenti, deve fare tendenza. Occorrono allora risorse per incentivare le aziende più innovative che, insieme al prodotto di qualità più alta, sappiano offrire strategie creative di distribuzione adeguata attraverso distribuzioni dirette ma anche distributori automatici che nel poco tempo, nei brevi intervalli scolastici, sfornino prodotti accattivanti ma buoni per la salute. Sarebbe in un solo colpo un beneficio alla salute di tanti e uno straordinario stimolo all'innovazione di prodotto di tante aziende di produttori. Sono altrettanto d'accordo però che accanto a questo ci sia bisogno di una nuova regolamentazione dei messaggi pubblicitari, un argine che contenga il danno. Ma dico di più: occorre una contro strategia mediatica. Se nella società della comunicazione il 70 per cento delle opinioni dei cittadini, nonché gli stili di vita, si formano sull'onda dei messaggi pubblicitari, occorrono risorse adeguate per una aggressiva, convincente strategia di *marketing* sociale pubblico; una strategia volta ad indirizzare comportamenti alimentari saggi perché qui il *business*, gli utili sono da distribuire tra tanti; sono di natura diversa dai soldi, investono standard del benessere psicofisico che si possono misurare in più concentrazione, più efficienza nello studio, nel lavoro, più consapevolezza di tipo salutistico ma anche sociale, e anche maggiore salvaguardia della biodiversità. Allora così tanti utili in prospettiva meritano un *marketing* pubblico delicato. Voglio considerare queste mozioni non un auspicio generico ma la base da cui partire per azioni concrete; un impegno del Governo sulle questioni poste. Mi accontento di un inizio di un impegno concreto.

Nella nostra esperienza credo ci siano il gioco e la corsa, che però oggi diventano difficili non soltanto per un difetto di educazione ma per l'impossibilità di usufruire di spazi,

Nel 2005 - ne hanno riportato notizia i giornali - è andato "in pensione" Günter Euringer, il bambino simbolo della barretta al cioccolato, che nel 1970 correva a perdifiato

Mi avvio ad una rapida conclusione per fare tesoro di quanto è stato detto. Io penso che esista una necessità,

Ricordo che qualche anno fa nel gruppo *scout* di cui facevo parte accanto all'intangibile simbolo delle nostre radici, veniva messo un altro intangibile simbolo del nostro egoismo: era la fotografia di uno di quei bambini che hanno tanto campo davanti e nessun fiato per correre. Non si ottenne un grande risultato in termini di peso perduto, ma qualche *brioche* andò di traverso.

cari colleghi, come molti di voi hanno già detto recenti statistiche ci hanno fornito dati molto preoccupanti che indicano come l'Italia - di fatto - sia uno dei Paesi dell'Unione europea con il più alto numero di bambini in sovrappeso. Secondo una ricerca scientifica, denominata "Okkio alla salute", promossa dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel nostro Paese è in sovrappeso il 23,6 per cento dei bambini tra i sei e i dieci anni, mentre il tasso di obesità nella stessa fascia d'età arriva al d'età arriva al 12,3 per cento. Il che, tradotto, significa che più di un bambino su tre ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Riportando questi valori a tutta la popolazione di bambini di età compresa tra i sei e i dodici anni, si giunge ad una stima di più di un milione di bambini sovrappeso. Ebbene, in Italia questo è un problema che assumerà una rilevanza sociale sempre maggiore, visto che in Europa il sovrappeso in età scolare cresce al ritmo di circa 400.000 casi l'anno. Soffermiamoci per un attimo sulle problematiche connesse all'obesità: ad essa sono associate sia conseguenze precoci, ossia problemi di tipo respiratorio, articolare, nonché disturbi dell'apparato digerente o di carattere psicologico, sia conseguenze tardive, dal momento che l'obesità infantile è un fattore predittivo di obesità

si associno disfunzioni di natura cardiocircolatoria, muscoloscheletrica, metabolica e disturbi alimentari, fino ad arrivare allo sviluppo di tumori del tratto gastroenterico. A tale proposito, un dato su cui riflettere è che dal 30 al 60 per cento dei bambini obesi mantengono l'eccesso ponderale in età adulta. Inoltre, l'adulto che è obeso fin dall'età evolutiva avrà un maggiore rischio di mortalità e morbilità rispetto ad un suo pari che non era obeso quando era bambino. Cerchiamo ora di analizzare le radici del problema. A parte i rari casi di obesità legati ad alterazioni ormonali quali ipotiroidismo o disfunzioni surrenali, essa è la diretta conseguenza di una eccessiva e/o cattiva alimentazione, legata o meno ad una ridotta attività fisica e a fattori di tipo genetico e familiare. Quindi, familiarità, sedentarietà e *status* economico, connesso spesso al livello di istruzione soprattutto della madre. Da ciò si deduce in primo luogo che è necessario educare le madri, affinché possano poi educare - a loro volta - i figli. In che modo? piuttosto - le loro scelte verso alimenti sani e nutrienti. Non c'è dubbio che un bambino che impara a mangiare le merendine continuerà a protrarre queste cattive abitudini anche da adulto; impara a mangiare la frutta manterrà queste buone abitudini anche da adulto. Quindi, sono importantissimi i primi anni di vita dei nostri bambini.

cui più frequentemente si presenta l'obesità infantile. Credo che così come appare chiaro che la prevenzione dell'obesità infantile passa attraverso un'alimentazione varia ed equilibrata, non deve essere sottovalutata l'importanza di una regolare attività fisica. In altre parole, è necessario utilizzare tutti i mezzi a disposizione per promuovere e consolidare nuovi stili di vita, che rappresentano la base

ricordato in Commissione sanità) una notevole riduzione di spesa per quanto riguarda la sanità. Bisogna soffermare l'attenzione sull'adozione di strumenti di sensibilizzazione che, attraverso la comunicazione istituzionale, possano promuovere un nuovo approccio al problema. Ed in quest'ottica non si può sottovalutare il ruolo della televisione, che spesso agisce negativamente attraverso la pubblicizzazione di merendine e *snack* (di solito tutti alimenti ipercalorici), molto spesso proprio durante le trasmissioni che interessano i bambini. In Italia, gli *spot* che pubblicizzano alimenti ricchi di zuccheri, grassi e sali interessano il 36 per cento della pubblicità e - ovviamente - nessuno di essi ammonisce circa il corretto consumo di tali cibi. Questi dati indicano la necessità di un sistema di limitazioni normative per la pubblicità commerciale, che protegga i minori dagli effetti dannosi e - nello steso tempo - valorizzi la produzione di qualità. A tale scopo, però, è necessaria anche la collaborazione della grande e media distribuzione, che deve definire regole deontologiche per introdurre per introdurre il criterio della qualità nutrizionale fra le scelte che presiedono alla definizione del valore della vendita. media ma anche e soprattutto scuola, perché nutrirsi bene deve essere considerato come uno dei primi insegnamenti da dare ai nostri bambini. Trovo che l'ora di ginnastica

l'educazione fisica e lo sport. Chiedo a tutti noi se questi spazi sono presenti oggi in tutte le scuole italiane, o se anche in questo senso non ci sia una disparità tra scuole private e pubbliche o tra scuole del Nord o del Sud. Questo è l'appello che rivolgo oggi al Governo. Credo che sia anche fondamentale introdurre

ecologiche, messe in stretto contatto con le scuole, in cui i bambini si recheranno per imparare come si mangia, cosa sono i cibi e quali sono i valori nutrizionali. Su questa spinta dovrebbero nascere tante altre del genere in Italia, non lasciati alla volontà dei singoli dirigenti scolastici. Sempre nell'ambito scolastico deve partire una rivalutazione del consumo di acqua e frutta, quest'ultima da sostituire a pizzette e patatine durante la ricreazione. Appare evidente come l'obesità infantile sia un problema complesso, che può portare con sé anche un grave disagio psicologico per il bambino: alla mancanza di autostima, tra l'altro, spesso si accompagna anche un disturbo del comportamento alimentare. Noi tutti sappiamo quanto oggi la la patologia legata al comportamento alimentare sia in grande aumento tra gli adolescenti italiani e non soltanto tra le femmine ma anche nei maschi. Da questo quadro si evince l'urgenza di un intervento coordinato e strutturale, proprio in considerazione dell'elevato costo sociale che il fenomeno sta assumendo per la popolazione italiana.

Le mozioni ci consentono oggi di affrontare il grave problema dell'obesità infantile, che ha assunto e può assumere connotati allarmanti per la salute dei giovani con evidenti problematiche sanitarie e sociali nell'età adulta. È una questione sociale di grande rilevanza, conseguenza di una società evoluta ed anche dei nostri stili di vita. Se in alcune parti del mondo la fame è un male che dilaga e miete vittime soprattutto in tenera età, nella nostra parte del pianeta si verifica invece il problema opposto. I bambini dell'Occidente aumentano invece di peso, con gravi conseguenze sulla loro salute ma anche sul loro stato psicologico.

È stato verificato, infatti, che i bambini in sovrappeso già a partire dalla scuola dell'infanzia mostrano maggiori sintomi di depressione, ansia e solitudine rispetto ai bambini normopeso e che questi sentimenti si intensificano poi negli anni. sovrappeso è considerata una condizione molto stigmatizzante e i soggetti che ne soffrono sono spesso colpevolizzati. L'esperienza di essere così stigmatizzati quasi sempre conduce poi a vissuti negativi proprio nel bambino. In Italia, poi, il messaggio pubblicitario è avvertito con grande enfasi e può modificare il nostro stile di vita e, quindi, incidere sulle abitudini alimentari delle categorie più sensibili, tra cui annovero proprio quella

sulle confezioni e che le scritte esaltano solo la presenza di vitamine e di ferro. Sappiamo benissimo, signor Presidente, che questi elementi nutrizionali sono molto marginali e che, di fatto, i prodotti contengono, invece, molti grassi.

In definitiva, credo che tutte le istituzioni debbano impegnarsi anche nei confronti di quei produttori che non utilizzano un messaggio pubblicitario corretto e veritiero e che, quindi, non si debbano avere remore a dare indicazioni ed informazioni, in tutte le forme

Ricordate le battute tipo "Cicciabomba cannoniere", che davano fastidio a tutti i bambini delle nostre classi quando venivano etichettati così? Immaginate l'autostima come viene a diminuire. Pensate poi che quel bambino all'80 per cento andrà incontro a problemi respiratori e renali

di solidarietà nei confronti nei nostri cittadini, ma anche in termini economici; la nostra sanità non può affrontare costi così elevati a fronte di messaggi

E mi stupisce che qualcuno abbia anche commentato in senso negativo ciò che si è fatto in California, dove il famoso Schwarzenegger ha deciso, criticato da tanti, di vietare la vendita nelle scuole di quelle bevande e di quelle merendine che oggi ritroviamo in ogni angolo delle nostre città, cercando di intervenire non vietando la pubblicità, non togliendo la libertà di promuovere i propri prodotti, ma vietando quel metodo subdolo di dare dei messaggi distorti, che inducono in maniera falsa a pensare di aiutare i nostri bambini

Nelle nostre scuole stiamo riempiendo di compiti e di nozionismi i nostri bambini e li teniamo incollati alle sedie senza farli muovere e senza far fare loro pratica sportiva. Abbiamo ancora scuole dove non sono praticabili le aule per fare un minimo di ginnastica, un minimo di movimento. Quindi, ha fatto bene il ministro Fazio a promuovere in Italia tutta una serie di iniziative che porteranno ad l'attività fisica e lo sport tra i giovani; ma non lo sport competitivo: lo sport amatoriale, quello che porta al movimento, quello che probabilmente è molto più efficace di tante medicine per prevenire le patologie. Ecco perché sono d'accordo con questa mozione e perché partecipo veramente con entusiasmo e parlo, lo ripeto, con il cuore. Stiamo facendo una scelta importantissima e, al di là delle parole, ciascuno di noi si deve sentire responsabilizzato a portare delle idee; ma non idee generiche, o che vadano a succhiare risorse senza di fatto risolvere problemi e senza nemmeno toccare la

la mia amata Sardegna, fortunatamente, è una delle regioni che subisce meno questo problema. Nel guardare i dati ho però visto che è la regione che invece sta andando più velocemente incontro ad un aumento degli obesi.

obesi andrà incontro alla obesità; non ci rendiamo conto, purtroppo, che le patologie legate alla obesità stanno aumentando e stanno facendo crescere i costi della sanità a livelli incredibili. Concludo cercando di fare riflessioni anche come medico.

È senz'altro necessario, come rappresentato dalle mozioni, che la promozione della salute inizi nell'ambito familiare affinché fin dall'infanzia si assumano stili di vita sani. La sana alimentazione è uno dei determinanti fondamentali per la tutela, la promozione e, ove necessario, il recupero della salute, per contrastare non solo l'obesità ma anche le patologie croniche ad essa associate, che hanno peraltro una ricaduta in termini di costo sociale che si avvicina a 30 milioni di euro l'anno, a causa della perdita di produttività, delle complicanze cliniche e delle cure correlate. È possibile evidenziare un quadro aggiornato del fenomeno sovrappeso ed obesità tra i bambini italiani grazie al progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età sei-diciassette anni: indagine Okkio alla salute", che il Ministero- Centro controllo malattie ha affidato all'Istituto superiore di sanità (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute). Il progetto, al quale hanno aderito tutte le Regioni, ha reso possibile, per la prima volta in Italia, con un'unica metodologia e su un campione rappresentativo di bambini della terza classe della scuola primaria (45.590 in 2.610 scuole), la raccolta dei dati concernenti peso e altezza (con il calcolo dell'indice di massa corporea), principali abitudini alimentari, attività fisica svolta e comportamenti sedentari. I dati hanno fatto emergere una prevalenza molto elevata di sovrappeso ed obesità, con notevoli differenze tra le Regioni e la diffusione tra i bambini di abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e predispongono all'aumento di peso. È stata inoltre avviata anche la sorveglianza sugli stili di vita degli adolescenti attraverso l'*Health Behaviour in School-aged Children* uno studio multicentrico svolto in collaborazione con l'ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che consentirà di raccogliere dati con rappresentatività regionale. Questa seconda fase del progetto permetterà di acquisire informazioni sui comportamenti relativi alla salute in età pre-adolescenziale ossia in quella fascia di età nella quale si instaurano e si rafforzano molti comportamenti non salutari: alimentazione scorretta, ridotta attività fisica, iniziazione al fumo e consumo di alcool. Sono necessari interventi intersettoriali con il coinvolgimento sia delle istituzioni centrali e locali, appartenenti a settori diversi da quello sanitario, sia della società civile intesa come sistema produttivo, associazionismo, volontariato, nell'ottica della «salute in tutte le politiche», approccio strategico sostenuto sia dall'Unione europea che dall'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo le indicazioni dell'Unione Europea e, in particolare, dell'Organizzazione mondiale della sanità, è stato approvato il programma nazionale «Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari», una strategia globale per contrastare i quattro principali fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili (fumo, abuso di alcool, dieta scorretta e inattività fisica)

l'obiettivo è, quindi, adottare una strategia volta a facilitare scelte e comportamenti adeguati attraverso l'informazione e una idonea impostazione delle azioni regolatorie, senza condizionare direttamente le scelte individuali, ma adottando politiche di collettività che possano ad esempio favorire lo sviluppo di un ambiente urbano che incoraggi l'attività fisica o di un sistema di distribuzione che favorisca i consumi di frutta e verdura. È essenziale: *a)* promuovere comportamenti salutari attraverso varie iniziative come la promozione dell'allattamento al seno. La tutela dell'allattamento al seno e una corretta informazione sull'alimentazione dell'infanzia rappresentano un argomento al quale questo Ministero ha prestato, da sempre, la massima attenzione. In questo ambito è stato elaborato il documento "Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno", che rappresenta la *policy* nazionale sulle problematiche connesse all'allattamento al seno e ai sostituti del latte materno. Inoltre, è stato istituito il "Comitato nazionale per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno", finalizzato all'implementazione di una rete nazionale su questa tematica; *b)*promuovere prodotti sani per scelte sane migliorando la composizione degli alimenti e sviluppando politiche agricole adeguate. Risulta fondamentale contribuire all'acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli in campo alimentare, far conoscere la qualità dei prodotti agroalimentari, riscoprire l'importanza del mangiare sano mediante un approccio a tutto campo e non impositivo, con una trattazione multidisciplinare e trasversale e con l'interessamento di tutti gli operatori del settore (produttori agricoli, trasformatori, addetti alla ristorazione, educatori, medici, eccetera) e di altri enti interessati (istituzioni centrali e locali, università, associazioni di consumatori, istituti di ricerca, Particolarmente efficace la valorizzazione del modello alimentare mediterraneo, la riscoperta di prodotti agroalimentari tipici del territorio, l'educazione alimentare intesa come un percorso formativo stabile per i ragazzi in età scolare, la qualificazione dei servizi di refezione collettiva. Il *target* privilegiato, rappresentato dai ragazzi in età scolare, va raggiunto attraverso percorsi didattici interattivi, sia in classe sia in attività esterne, che invitino i più giovani ad avere un rapporto positivo con il cibo, a riscoprire il gusto e le peculiarità del mondo rurale, a riconoscere la qualità. A tal fine, il protocollo d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siglato nel marzo 2008, si propone di realizzare interventi intersettoriali per sensibilizzare i consumatori, fin dal momento dell'acquisto dei prodotti, sull'importanza di una alimentazione equilibrata. L'intesa mira, inoltre, a valorizzare la dieta mediterranea, per i suoi effetti positivi sulla salute e quale stile di vita unico al mondo, e dedicare particolare attenzione all'alimentazione di alcuni gruppi di popolazione, caratterizzati da esigenze nutrizionali specifiche e per questo motivo più vulnerabili,

anche in ambienti come la scuola e i luoghi di lavoro; *c)*promuovere i consumi salutari e quindi educare al consumo consapevole. Tra le varie iniziative particolare importanza assume l'attivazione, nell'ambito dell'intesa sancita con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di progetti finalizzati ad educare i giovani, ad un consumo consapevole, ad una alimentazione equilibrata e a stili di vita corretti. Devono essere forniti agli insegnanti strumenti didattici, destinati ad elaborare percorsi formativi, e ad avviare un'azione di sensibilizzazione e informazione presso le famiglie. Tra le iniziative avviate, il progetto pilota "frutta snack" ha rappresentato un'esperienza di educazione alimentare, che nell'anno scolastico 2007-2008, ha coinvolto 80 scuole secondarie di secondo grado di Roma, Bologna e Bari, in collaborazione con aziende private del *vending* e della produzione ortofrutticola per incentivare il consumo di frutta e verdura tra i ragazzi. Tale progetto ha previsto non solo l'istallazione di distributori automatici di frutta fresca nelle scuole interessate, ma anche un programma di formazione/informazione dei docenti e iniziative di sensibilizzazione e comunicazione per le famiglie e gli studenti, nonché attività di monitoraggio e valutazione dei risultati. La necessità di sviluppare un approccio intersettoriale alla promozione della salute ha portato, nell'ambito di "guadagnare salute", alla istituzione nel 2007 della "Piattaforma nazionale sull'alimentazione, l'attività fisica e il tabagismo", quale sede d'incontro fra tutte le istituzioni, le associazioni e gli organismi interessati La piattaforma, di cui nella composizione modificata e aggiornata si è tenuta la seduta di insediamento nello scorso mese di novembre, vede la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle Regioni e Provincie autonome, delle associazioni di categoria della filiera alimentare e del commercio, delle associazioni dei consumatori, di istituti di ricerca, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti Proprio per la funzione di concertazione svolta dalla Piattaforma, sarà possibile continuare a sviluppare alcuni elementi caratterizzanti, il programma "Guadagnare salute": promozione della salute come bene pubblico; approccio trasversale ai fattori di rischio; definizione di strategie intersettoriali, tra loro coordinate; sviluppo di sinergie per i cittadini, per trasformare le buone pratiche in interventi consolidati; stipula di appositi protocolli di intesa tra il Ministero della salute, *leader* e promotore del programma, e gli altri soggetti coinvolti, ossia istituzioni centrali, rappresentanze della società civile e del mondo produttivo. Si è reso necessario avviare una serie complessa di attività, finalizzate alla modifica di abitudini alimentari scorrette ed alla promozione di una vita attiva, tramite intese siglate con i Ministri dell'istruzione, delle politiche giovanili e delle politiche agricole e forestali. *a)*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il MIUR ha sottolineato l'estrema attualità della nutrizione, della sicurezza alimentare, degli obblighi nazionali e comunitari rivolti alla migliore conoscenza dei vari aspetti sulla salute: tali tematiche devono costituire oggetto di attenzione e riflessione da parte di docenti e studenti in un'ottica interdisciplinare. Infatti, un ragazzo male alimentato rischia di diventare un adolescente insoddisfatto del proprio aspetto e della propria inefficienza, sino a divenire spesso un adulto malato, le cui cure ed i relativi costi ricadono sull'intera collettività. Ciò può essere fortemente limitato con una migliore conoscenza nutrizionale, con l'informazione agli studenti e con la formazione per i docenti e il personale scolastico. Dal corrente anno scolastico è stata avviata presso alcune istituzioni di livello primario la fase iniziale del Progetto "scuola e cibo" - piani di educazione scolastica alimentare. Si tratta di un'iniziativa di notevole rilevanza didattico-educativa che il MIUR intende progressivamente estendere su tutto il territorio nazionale e per tutti gli ordini di studio. Il Progetto è legato all'attualità dell'argomento alimentazione e all'assegnazione a Milano dell'EXPO Universale 2015 sui temi del cibo e della nutrizione. La prima fase è la realizzazione di un Progetto pilota da svolgersi nel corrente anno scolastico 2009-2010, testato su un campione di 15 scuole con circa 75 classi primarie (4a e 5a elementare) e che coinvolge circa 1.500 alunni complessivamente. In particolare, sono state coinvolte rispettivamente cinque scuole di Roma e provincia, di Milano e provincia e di Catania e provincia, ognuna, con 4-5 classi elementari diverse, oltre al personale docente interno ed esterno. Il Progetto diverrà operativo a livello nazionale nell'anno scolastico 2010-2011, ed è prevista l'adozione di un testo base sull'educazione alimentare. Il MIUR valuterà collaborazioni e sinergie nel settore, anche per operare in prospettiva del 150° anniversario dell'Unità d'Italia (2011) e dell'EXPO Universale 2015, nonché le possibili intese con le associazioni di categoria per rilanciare il *Made in Italy* del settore alimentare, anche in accordo con i comparti della ristorazione e del turismo. Con la diffusione del Progetto verrà realizzata ogni anno una "Giornata aperta" nelle scuole del territorio nazionale sulle tematiche cibo-acqua-mense scolastiche, in accordo con il Ministero degli affari esteri e la FAO. inoltre in corso di realizzazione la pubblicazione informativa "*Vademecum* sulla sicurezza e la qualità degli alimenti", in collaborazione con il Dipartimento della gioventù della Presidenza del consiglio dei ministri, che verrà gratuitamente distribuita nelle scuole secondarie nazionali di primo grado. Infine, si segnala la partecipazione al programma comunitario «Frutta nelle scuole», che nel nostro Paese si realizza con l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tale programma si propone di far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini, aumentandone la porzione giornaliera nella loro dieta nella fascia di età in cui si formano le abitudini alimentari. Attivato a partire dall'anno scolastico 2009-2010, per la prima annualità vedrà il coinvolgimento di circa 800.000 bambini delle scuole primarie (circa un terzo della popolazione scolastica primaria) e, nello specifico, si articolerà nella distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi, nel rispetto della stagionalità e territorialità, privilegiando prodotti di qualità certificati e prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata certificata. Al fine di rendere efficace e sostenibile il programma, si prevede la realizzazione di misure di accompagnamento nell'ambito di quelle suggerite dall'Unione europea, quali attività di informazione e sensibilizzazione per i docenti e i genitori e iniziative per far conoscere e scoprire i prodotti ortofrutticoli ai più giovani e prolungarne l'effetto di induzione del consumo. Il principale obiettivo dell'Accordo sui rischi comportamentali in età 6-17 anni è la sensibilizzazione, in particolare dei giovani, ma anche della popolazione generale (comprese le persone diversamente abili e quelle portatrici di disagio psichico o disturbo mentale) sull'importanza di uno stile di vita attivo, associato ad una corretta alimentazione. L'intesa promuove, inoltre, la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare per favorire fra i giovani un rapporto equilibrato con l'immagine corporea e contrastare quei fattori, socio-culturali presenti nell'insorgenza e nella diffusione di alcuni disturbi (anoressia, bulimia, obesità

un progetto per la promozione dell'attività motoria attraverso programmi basati principalmente sulle attività della vita quotidiana, (camminare, andare in bicicletta, fare le scale); queste attività, infatti, non richiedono molto tempo, sono svincolate dalla disponibilità di strutture, hanno costi molto contenuti e sono quindi accessibili anche alle fasce sociali svantaggiate. Ci si propone di sperimentare in cinque Regioni (Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia con il coordinamento della Regione Veneto-ULSS 20 di Verona), iniziative rivolte a tutta la popolazione, per facilitare lo sviluppo di reti locali di soggetti che concorrano alla promozione dell'attività motoria (associazioni, Comuni, scuole, operatori sanitari, educatori, istruttori e altri soggetti pubblici e privati), con il coinvolgimento strutturato dei medici di medicina generale. La comunicazione. Lo sviluppo di attività di comunicazione costituisce parte strutturale del programma "Guadagnare salute" ed è indispensabile strumento di informazione e promozione della salute; l'obiettivo delle iniziative di comunicazione rivolte alla popolazione generale e a gruppi specifici sarà la conoscenza dei comportamenti da adottare e delle opportunità offerte dal contesto socio-ambientale Anche per quanto riguarda le iniziative di comunicazione, la sinergia tra i diversi soggetti è elemento di fondamentale importanza per dare maggiore credibilità ai messaggi da veicolare e assicurare un'informazione univoca

per l'infanzia". Proprio in questi ultimi giorni è stato presentato ufficialmente il "Codice deontologico dell'Associazione italiana industria e prodotti alimentari (AIIPA), sezione prodotti per l'infanzia" concernente le problematiche relative alla primissima età, recependo così i contenuti del Decreto 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della Direttiva comunitaria n. 141 del 2006 sui sostituti del latte materno e le formule di proseguimento. Il Codice si pone l'obiettivo di contribuire ad assicurare ai lattanti e ai bambini una nutrizione sicura ed adeguata, proteggendo, promuovendo e sostenendo l'allattamento al seno, assicurando l'utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessario, sulla base di informazioni adeguate ed attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione. Gli orientamenti del Governo per le nostre imprese sono ispirati a principi di rigore e di sostegno, esplicitando al consumatore le buone pratiche produttive, il sistema dei valori e il modo di essere e di agire delle imprese interessate e prevedendo, nel contempo, per le aziende un valore aggiunto di rilevante importanza che obbliga ad un determinato standard di qualità. Con gli accordi stipulati nell'ambito di «Guadagnare salute» le organizzazioni più rappresentative del mondo delle imprese e dell'associazionismo hanno assunto un ruolo attivo nella promozione della salute, che le impegna, che le impegna, in particolare a sviluppare la ricerca tecnologica per le innovazioni di prodotto e di processo utili a migliorare la composizione degli alimenti, con la riduzione dei contenuti di zucchero, grassi e sale; migliorare la qualità dell'informazione pubblicitaria diretta ai consumatori, in particolare ai bambini ed agli adolescenti; fornire ai consumatori informazioni dettagliate sugli alimenti, tramite anche un'etichettatura completa e facilmente comprensibile. Sulla base di queste considerazioni, il Governo esprime consenso alle mozioni presentate.

il tema in esame è di interesse di tutti, le argomentazioni portate dalle mozioni presentate sono ampiamente condivisibili e, pertanto, anche il nostro voto sarà favorevole sui tre testi. Ciò che mi preme sottolineare con forza è in primo luogo la necessità che quanto si chiede di porre in essere con queste mozioni non resti una mera petizione di principio. È essenziale che si mettano a disposizione tutti gli strumenti necessari all'attuazione di quelle iniziative concrete che servono ad indirizzare i nostri bambini verso una buona educazione alimentare che permetta loro di non compromettere la salute in un'età così importante come quella della crescita. Abbiamo detto anzitutto che il primo ruolo educativo spetta ai genitori che, a volte, per una comprensibile affettuosa complicità, sono portati a cercare di soddisfare i desideri dei propri figli e che vanno invece informati di quali siano i rischi cui possono esporre i propri figli se indulgono eccessivamente in una alimentazione non equilibrata. In secondo luogo abbiamo evidenziato l'importanza della scuola. Su questo punto va sottolineata in particolare la necessità che vengano effettivamente messi a disposizione i fondi occorrenti per la messa in opera di iniziative volte all'educazione alimentare, ad uno stile di vita sano ed alla cura della propria salute. la necessità di una regolamentazione per quanto riguarda i messaggi pubblicitari rivolti ai più piccoli. Badate bene, nessuno vuole limitare la libertà di mercato e sappiamo che, come si dice, «la pubblicità è l'anima del commercio». Ciò che sembra doveroso è cercare di limitare in determinate fasce di programmazione il bombardamento pubblicitario con *spot* aventi ad oggetto determinati alimenti. È una misura semplice, già adottata in altri Paesi europei, che ha dato positivi risultati. Nel ribadire il nostro voto favorevole, voglio ancora una volta sottolineare come solo con la collaborazione di tutti i soggetti interessati saremo davvero in grado di preservare la salute dei nostri bambini e ragazzi, e quindi degli uomini di domani. Signor Presidente, colleghi, ci risulta facilmente condivisibile il fatto che l'obesità infantile sia un grave problema, non solo nel nostro Paese, ma a livello mondiale, come emerso emerso dagli autorevoli interventi che hanno animato la discussione sull'argomento. Maggiormente colpite sono le popolazioni dei Paesi occidentali, e l'Italia vanta purtroppo, all'interno dell'Unione europea, questo triste primato: siamo

Blair, che promosse una forte campagna di sensibilizzazione nelle scuole imperniata sulla dieta mediterranea. L'hanno fatto gli inglesi: a maggior ragione dobbiamo e possiamo farlo noi nel nostro Paese, noi che la dieta mediterranea la promuoviamo,

In conclusione, credo sia paradossale che in un Paese che vanta una ineguagliabile tradizione culinaria, un Paese ricco di ogni varietà di alimenti vegetali e animali, non riusciamo a conquistare la generazione dei più piccoli, sono invece catturati da messaggi pubblicitari di massa che rischiano assolutamente di standardizzare i consumi alimentari. Stiamo perdendo nel nostro Paese la cultura della cucina, che non è fatta solo di cibo ma anche di valori simbolici, quali sicuramente la convivialità,

Dobbiamo riscoprire il gusto e il tempo di mangiare a tavola tutti insieme, genitori e figli, con cibi possibilmente semplici e genuini. Per tutti questi motivi sosteniamo con convinzione gli impegni contenuti in tutte le mozioni in esame, non solo in quella presentata dal nostro Gruppo, auspicando che attraverso un auspicando che attraverso un piccolo, ma potenziale e molto efficace strumento di comunicazione istituzionale sia possibile riscoprire quella cultura dell'alimentazione che è sinonimo di un approccio sicuramente sano ed equilibrato al cibo fin dalla prima infanzia. Signor Presidente, vorrei riprendere solo alcuni degli argomenti che sono stati al centro del dibattito di questa mattina

obese, il doppio rispetto a cinque anni fa. Per questo gli stessi medici hanno lanciato una campagna contro l'obesità per il 2010. L'obesità crescente non è solo un problema italiano: è un fenomeno internazionale, al punto che l'Organizzazione mondiale della sanità, Ufficio regionale per ha tenuto ad Istanbul nel 2006 una conferenza ministeriale intergovernativa proprio per definire le strategie di contrasto al fenomeno in questione.

cure richieste proprio per le malattie associate all'obesità. Questa battaglia contro l'obesità è partita nel 2007 con un'iniziativa del Ministero della salute, che istituì allora un tavolo tecnico - ricordato anche dal sottosegretario Scotti composto dalle amministrazioni centrali, dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle associazioni di categoria della filiera alimentare e dei consumatori dalle organizzazioni sindacali, proprio per elaborare questa piattaforma nazionale sui temi dell'alimentazione, dell'attività fisica e del tabagismo. L'obesità, infatti, non è solo un problema estetico, ma porta con sé rischi per la salute ed è una delle prime cause del diabete, come abbiamo ricordato in quest'Aula qualche settimana qualche settimana fa; essa moltiplica i rischi di malattie cardiovascolari e può favorire alcuni tipi di tumore. Inoltre, è anche una fonte di disagio e di sofferenze psicologiche. Vorrei ricordare, a questo proposito, che anche se dobbiamo combattere il fenomeno dell'obesità, non possiamo però accettare la demonizzazione e la colpevolizzazione di chi soffre di questo problema. Vorrei ricordare che esiste anche uno stigma che, soprattutto tra i bambini, diventa escludente e va combattuto: spesso i bambini obesi sono oggetto di atti di bullismo, di violenza, di emarginazione nella scuola e tra i compagni di gioco. Gli obesi sono anche le vittime più evidenti, purtroppo, di un sistema sociale che da una parte ci vuole tutti magri - anzi più che magri, qualche volta anoressici, come appare dai modelli della pubblicità - e dall'altra esalta un consumo senza regole e senza limiti, in particolare del cibo. Per queste ragioni occorre sviluppare una maggiore consapevolezza anche circa l'influenza dei *media* sui comportamenti alimentari dei bambini e degli adolescenti. Vorrei ricordare, come sottolineava anche la senatrice Serafini, che in alcuni Pesi europei esistono delle normative che limitano la pubblicità delle normative che limitano la pubblicità commerciale in ordine all'alimentazione e al consumo. Tra i molti punti trattati nelle mozioni, in particolare nella nostra, vorrei ricordare l'importanza di prevenire l'obesità coinvolgendo le future madri e, io aggiungo, i futuri padri. Far crescere la consapevolezza nelle donne in gravidanza che un'alimentazione equilibrata, una regolare attività fisica e l'eliminazione di alcool e fumo possono aiutare la crescita sana del feto, e quindi del futuro bambino, è importante per cominciare ad educare anche i futuri genitori ad una capacità di sviluppare l'azione educativa con stili di vita che, partendo dal padre e dalla madre, siano un modello educativo per Per fare ciò occorre però creare una rete di servizi, bisogna supportare i nuovi genitori anche dopo la nascita del bambino, almeno nel primo anno di vita, non solo per affrontare problemi come la depressione dopo la gravidanza, ma anche per aiutare a far crescere meglio il bambino. Quando poi il bambino potrà ci auguriamo - frequentare il nido, la scuola per l'infanzia, la scuola elementare, si renderà necessaria una collaborazione tra scuola e famiglia. Vorrei qui ricordare come sia difficile molte volte costruire una collaborazione tra scuola e famiglia per favorire un'alimentazione equilibrata, che riduca l'eccesso di grassi e di zuccheri che sempre più fanno parte di prodotti di largo consumo quotidiano. perché spesso oggi i genitori chiedono al servizio di refezione e a chi lo gestisce (gli enti locali) di adeguarsi ai gusti dei bambini e non di educare i bambini e di autoeducare in qualche modo anche la famiglia ad una corretta alimentazione. Quindi, c'è da affrontare sul territorio questo tema. Infine, l'attività fisica: se ne è parlato, purtroppo però non ci sono più spazi per i bambini. Dobbiamo prenderne atto: gli spazi per giocare nei cortili cortili o nelle scuole sono ormai ridotti al lumicino. I cortili sono diventati dei parcheggi; molto spesso gli spazi nelle scuole sono serviti per ampliare altri tipi di attività; in una società che invecchia i bambini danno fastidio se giocano sotto casa; i giardini non sono sicuri. Quindi, i nostri bambini passano il tempo davanti alla televisione e al computer, aumentando non solo il loro peso, ma anche la loro solitudine. Lo sport nella scuola non si fa,

a sostenere finanziariamente e con spazi adeguati l'attività delle società sportive che si rivolgono in particolare ai bambini. Mi fa piacere leggere in un comunicato stampa che il ministro Fazio intende inserire l'attività fisica

la prego di concludere.

un intervento concreto e soprattutto che nasca dall'allarme che noi avvertiamo per ciò che sta accadendo nel mondo. Nel mondo - lo abbiamo detto questa mattina - l'obesità infantile sta crescendo a dismisura;

quelle cardiorespiratorie o infettive o a patologie quali il diabete che - ne abbiamo parlato nei giorni scorsi - è una malattia drammatica per come si sta sviluppando. - se mi permettete - anche a grossi problemi psicologici: abbiamo parlato anche del fatto che, purtroppo, i bambini obesi molte volte diventano il bersaglio del bullismo, sono bambini che vanno incontro ad una disistima e quindi a problemi che si ripeteranno anche nel futuro e che lasceranno degli strascichi

che sradichino certi costumi presenti in un Paese come il nostro che, per assurdo, sta promuovendo la cultura dell'alimentazione americana che tanti drammi ha creato in America, con una crescita a dismisura di paninoteche ma soprattutto di hamburgherie. a danno della nostra storia agroalimentare, della nostra produzione. Vi ho raccontato della mia magnifica Sardegna, dove crescono le hamburgherie e i nostri prodotti agroalimentari, che sono meravigliosi, che sono il nostro vanto, che sono veramente naturali e sarebbero l'alimentazione eccellente per i bambini, vanno invece a marcire perché non trovano mercato soprattutto interno. Ecco perché ciò che ha detto il sottosegretario mi induce ad un moderato ottimismo. Sono sicuro che il Governo Berlusconi stia portando avanti delle ottime iniziative. Ricordo quella quella che ci è stata presentata nei giorni scorsi dal ministro Fazio per incentivare l'attività fisica nei giovani, soprattutto nelle scuole. L'attività fisica, non lo sport competitivo. L'attività fisica che sta venendo a mancare, la cosa essenziale, il movimento, che è la vera cura per i nostri bambini.

sociali, alimentari, storici, culturali. Come facciamo nella scuola a chiedere che si possano informare i nostri giovani sulla cattiva alimentazione se contemporaneamente non tracciamo dei percorsi didattici e non offriamo strumenti per poter intervenire? Come possiamo pensare che possano cambiare la propria alimentazione i bambini, benché ben informati a scuola, se non insegniamo ai genitori a portare essi per primi uno stile di vita nella propria famiglia? Io sarò Io sarò uno dei primi a dover essere coerente con quanto dichiaro. Ecco perché credo che tutte le proposte che sono state presentate dal Sottosegretario dovranno essere moltiplicate. Il *target* della scuola

di legge estremamente interessanti, di poter aggiungere la mia firma. Naturalmente spero che su una battaglia così importante, così urgente per il futuro della nostra Nazione non ci siano divisioni tra maggioranza e minoranza o una gara tra chi è più bravo o chi fa le proposte migliori:

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

la mozione nasce da una convergente presa di coscienza da parte di tutti i Gruppi politici del Senato della necessità di indirizzare, stimolare, sostenere politicamente ed anche impegnare il Governo a svolgere un'intensa attività diplomatica in ambito internazionale per dare sviluppo positivo a tutte le iniziative che tendono a ridurre la presenza degli ordigni nucleari, sino a giungere ad una loro completa eliminazione.

stessi otto grandi Paesi a svolgere un'attività intensa ed efficace, proprio perché si considera la presenza degli ordigni un autentico pericolo per l'umanità.

per la non proliferazione degli ordigni tendente poi a raggiungere l'annullamento della presenza degli stessi. Nel frattempo, la Federazione russa e

possesso. Gli Stati Uniti hanno poi convocato per la prossima primavera un vertice sulla sicurezza nucleare, al quale hanno invitato anche l'Italia.

miliare sulla quale costruire il processo efficace ed effettivo di non proliferazione.

un quantitativo di ordigni nucleari assolutamente inutile, assolutamente non rispondente a reali esigenze di deterrenza o di impiego operativo. Abbiamo - stupidamente una massa di ordigni nucleari che non rappresentano altro se non un pericolo per un possibile lancio inavvertito, remoto ma possibile, e soprattutto per una proliferazione degli stessi ordigni. Chiunque ha nozione e coscienza di che cosa vuol dire un'esplosione nucleare (cosa di cui tutti si riempiono la bocca non sapendo neanche di che cosa si tratti), chiunque ha coscienza di che cosa succederebbe se, anche in termini di deterrenza, uno Stato desse il via ad un'esplosione nucleare, si rende conto che disporre di migliaia di ordigni nucleari è stupido, è ridicolo,

se si corrono i rischi che prima ho ricordato, se ne corre anche un altro, estremamente pericoloso, e cioè che il terrorismo venga in possesso di un ordigno nucleare, nel qual caso tutti i freni a cui si può fare riferimento per un comportamento comunque equilibrato da parte dei Capi di Governo (anche dei Governi meno affidabili) verrebbero meno, in quanto il terrorismo ha dimostrato di non avere nessuno scrupolo nell'usare qualsiasi mezzo pur di colpire l'avversario. Fatte queste osservazioni, considerato che la stessa Unione europea ha messo a punto una direttiva per

ed il Governo italiani hanno effettivamente capito l'importanza di impegnarsi per eliminare ogni forma di proliferazione. La impegna quindi il Governo ad intraprendere ogni possibile iniziativa sul piano diplomatico per promuovere la sicurezza attraverso il rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione e disarmo, avendo a mente la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e gli impegni assunti nel quadro del G8 con la Dichiarazione dell'Aquila Governo per rafforzare, in vista della Conferenza di riesame del 2010, il Trattato di non proliferazione nucleare (che, come ho detto prima, rappresenta la pietra miliare per l'avvio di un'efficace azione di disarmo), nonché per la tutela dell'impiego pacifico dell'energia nucleare. a sostenere un processo di disarmo nucleare di non proliferazione, propiziando l'entrata in vigore del Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari

impegna inoltre il Governo a promuovere ulteriori riduzioni delle testate nucleari esistenti, fino a giungere alla loro totale eliminazione, attraverso contatti diretti (qui vi è un grande spazio

perseguire l'obiettivo della prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio extraatmosferico, proteggendo tutto il sistema satellitare, che condiziona ogni giorno di più, non solo l'attività di informazione in ambito mondiale, ma anche tutta una serie di altre attività svolte a tutela della società umana. Infine, la mozione esorta il nostro Governo ad assumere attività e iniziative per contribuire a risolvere alcuni problemi delicati e nevralgici, come quello relativo al Medio Oriente, anche in relazione alla possibilità o meno per l'Iran di costruirsi un ordigno nucleare. Queste sono, da una parte, le ragioni che hanno mosso la presentazione della mia mozione e, dall'altra, specificamente gli impegni che vengono richiesti al Governo, che mi auguro vorrà accettare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

come l'Italia possa contribuire a rafforzare un'azione internazionale perché la minaccia nucleare non solo non aumenti ma possa finalmente concludersi. Stiamo facendo

notevole a questa mozione perché si tratta di un atto politico importante. Tante sono le mozioni importanti, ma il fatto che tutti i Capigruppo ne sottoscrivano una è una indicazione politica fondamentale, che credo che credo esprima un elemento importante che la politica non deve sottovalutare. Non dobbiamo pensare che battaglie ideali, anche difficili, non debbano avere la giusta forza per essere portate avanti. avanti. Sembra che le decisioni dei consessi internazionali siano in qualche modo soltanto carta o un richiamo alle buone intenzioni, e che poi

di idealità o di mettere insieme buone intenzioni. Siamo di fronte ad uno dei punti fondamentali della sicurezza del mondo. È davvero un fatto

politica precisa. Quel Consiglio di Sicurezza che discuteva proprio di questo tema, quello che ha prodotto la risoluzione n. 1887 sul disarmo nucleare.

un segnale importante, ed è giusto che l'Italia su questo, con tutta la forza che può imprimere, dia una mano affinché detto processo vada avanti, lo faccia sentire come qualcosa di fondamentale e importante.

per quanto riguarda il nuovo accordo sulla riduzione delle armi strategiche. Ricordiamo tutti che nell'ultima fase della Presidenza Bush vi fu un momento di tensione abbastanza forte tra gli Stati Uniti e la Russia,

considerare con attenzione quelle che sono le potenze e far sì che il lavoro diplomatico impedisca decisioni politiche che possono rendere più difficile il dialogo e la possibilità di arrivare ad accordi. Con la decisione di Obama di tornare indietro rispetto a quella proposta di scudo, si è riaperto invece un dialogo con la Russia, che ha portato a quell'atto, sicuramente importante. Il mondo, che era riuscito, nei nei momenti in cui si cominciava ad utilizzare il nucleare e l'atomica - con i disastri che il senatore Ramponi ha prima descritto - a darsi delle regole per contenere questo tipo di minaccia,

Stati che non hanno sottoscritto il Trattato di non proliferazione possono in qualche modo avanzare rispetto a questi percorsi e il fatto che noi sappiamo che esiste un terrorismo internazionale che potrebbe - Dio ce ne scampi e liberi: speriamo non avvenga mai! - entrare in possesso di armi di questo tipo ci rende tutti ancora più responsabili. È chiaro che, per deprecare l'azione della Corea del Nord che, nonostante le pressioni della comunità internazionale, è andata avanti sul proprio programma nucleare, per fermare la volontà iraniana - se questa è - di andare avanti con il proprio programma, c'è bisogno di cominciare con atti importanti che dimostrino che già in casa nostra, nell'ambito cioè delle nostre possibilità, queste decisioni le assumiamo. Il fatto che intanto si decida, ciascuno nelle proprie competenze, ma in consessi internazionali che poi impegnano i diversi Stati, a ridurre complessivamente gli armamenti nucleari, credo sia importante e propedeutico per poter essere anche più forti nelle sanzioni verso quei Paesi che

questa azione diventa semplicemente un'azione di conoscenza, di messa in evidenza di problemi, senza però essere incisiva. Questo è un punto importante,

il punto è condiviso, e ricordo soltanto (perché è una discussione che abbiamo fatto, anche recentemente, nelle Commissioni esteri e difesa di Camera e Senato: nel momento in cui abbiamo parlato di Afghanistan, ad esempio), nell'attuale situazione di crisi internazionale, l'importanza che

evitare la proliferazione delle armi nucleari (ed ho detto al riguardo che spetta anche ai Paesi che le possiedono, pur avendo sottoscritto il Trattato di non proliferazione, promuovere il disarmo, perché è un messaggio che sta insieme);

e ovviamente - non perdiamo di vista quello che è un rischio che purtroppo esiste oggi per la sicurezza del mondo - scongiurare il terrorismo nucleare. Per tutte queste

di legislatura il Senato si è espresso molto compattamente per dire no alle *cluster bomb*, credo che sia un segnale bello e importante per l'opinione pubblica che il Senato in questa giornata sia impegnato in una discussione che vede tutti concordi e che dice al Governo italiano, all'Italia e a tutte le forze politiche: non consideriamo questo un obiettivo idealistico, pensiamo che possa essere un obiettivo perseguibile su cui lavorare con serietà e attenzione, non parlandone soltanto nei casi in cui se ne deve discutere perché la mozione viene presentata, non solo nei periodi natalizi in cui siamo tutti più buoni, ma facendolo diventare uno degli argomenti dell'agenda politica del nostro Paese all'ordine del giorno tutti i giorni.

anche in quella sede è stato presentato e approvato all'unanimità un rapporto sulla non proliferazione delle armi nucleari. Questo conferma che il nostro relatore e gli altri firmatari della mozione hanno fornendo una testimonianza concreta nel momento in cui il dibattito, a livello europeo ma anche mondiale, si sta sviluppando. A Parigi in quella sede fu anche fatto uno *screening* molto severo e preoccupato dei Paesi che dispongono oggi di testate nucleari o che sono impegnati nella ricerca nucleare: accanto a Paesi tradizionalmente riconosciuti, come Stati Uniti, Russia, Francia e Regno Unito, per i quali francamente non nutriamo grandi motivi

detentori di testate nucleari, ma sicuramente per motivi meno rassicuranti, per non dire decisamente inquietanti. Oltre alla non appartenenza ad alcuna intesa o Trattato di non proliferazione, allo START o ad altri accordi, c'è la loro palese indisponibilità ad accettare qualsiasi proposta di dialogo ma, soprattutto, a non tenere in alcuna considerazione le finalità ispettive dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, chiudendo la porte, non solo dei loro arsenali militari, ma anche delle centrali nelle quali si dovrebbe produrre solo energia a scopi civili. Occorre quindi rilanciare su scala mondiale - come ha detto il nostro relatore - un'azione di coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti i Paesi, partendo proprio dalla dichiarazione di non proliferazione adottata all'Aquila in occasione del G8 italiano,

sicuramente la Conferenza per il riesame del Trattato di non proliferazione, prevista per il prossimo mese di maggio, e il vertice sulla sicurezza nucleare, promosso dagli Stati Uniti per il mese di aprile. In queste due sedi occorrerà forse innescare una marcia in più, svolgere un'azione più incisiva, affrontando con coraggio proprio il tema dei Paesi che detengono testate nucleari ma che non riconoscono alcun trattato. Non so con quali parole si potrà inaugurare

sull'operato di alcuni Paesi membri dei vari trattati che riconoscono il Trattato di non proliferazione nucleare, ma che svolgono attività non del tutto trasparente di proliferazione: questo vale non solo per iniziative di ricerca o di produzione di energia nucleare a scopi civili, ma anche per azioni evidenti di implementazione mascherata di arsenali militari. Ci si chiede a quale scopo, se il nostro relatore, che è anche uomo competente per professionalità già dimostrate nella sua vita precedente a quella di politico, ha definito stupidi questi arsenali e ha detto che proprio non sappiamo che utilizzo che utilizzo se ne possa fare. Io da civile mi auguro che si possa immaginare uno smantellamento di queste testate e un utilizzo dell'energia che contengono a scopi civili. Nonostante i progressi di questi ultimi anni che hanno portato alla riduzione delle categorie di armamenti, l'obiettivo di arrivare ad uno smantellamento totale rimane, come si legge anche nella mozione, una vera e proprio utopia. La stessa mozione dice testualmente che sulla terra c'è un enorme numero di testate nucleari. È davvero preoccupante questa immagine, soprattutto per le ipotesi già ricordate di un errore umano e di un utilizzo da parte di organizzazioni terroristiche. Non vogliamo nemmeno immaginare che tipo di effetti produrrebbe un uso di questo tipo. È stato ricordato ‑ avevo la fortuna di essere al Parlamento europeo nel 2003 ‑ che nel secondo semestre della Presidenza italiana fu varata un'azione molto condivisa e convincente per la non proliferazione.

la mozione in discussione costituisce un'importante manifestazione di attenzione da parte del Parlamento su un tema di portata universale sul quale il nostro Paese, anche avvalendosi dell'opera di stimolo e sostegno proveniente dalle forze politiche, può continuare a svolgere un ruolo propositivo e di avanguardia negli anni a venire. Il fatto che essa sia stata sottoscritta dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari del Senato rappresenta sotto questo profilo un dato importante perché attesta un comune sentire delle forze politiche su questo importantissimo tema. La diffusione delle armi di distruzione di massa rappresenta una minaccia crescente per la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto alla proliferazione è diventato una crescente priorità dell'agenda internazionale, come dimostrato anche dalla particolare attenzione personale dedicatagli dal presidente statunitense Obama. L'impegno nel disarmo e nella non proliferazione rappresenta un elemento qualificante della politica estera dall'Italia e si basa su un ampio sostegno del Parlamento e della società civile. È un terreno che vede l'Italia tradizionalmente attiva su più fronti (alle Nazioni Unite, all'Unione europea, al G8 e nei processi di riesame delle maggiori convenzioni internazionali in primo luogo, nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nonché sul piano bilaterale con i nostri principali partner). Già durante la Presidenza italiana dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003 su nostro decisivo impulso era stata adottata la strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. In essa viene riconosciuta una responsabilità comune dell'Unione europea e degli Stati membri nell'affrontare i rischi legati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e nell'impegnarsi concretamente contro la loro diffusione; un impegno da portare avanti attraverso il rafforzamento del sistema internazionale di non proliferazione, la promozione dell'universalità degli accordi internazionali, la garanzia dell'attuazione e del rispetto dei rilevanti obblighi internazionali. Questi stessi principi sono stati alla base dell'azione italiana in ambito G8, durante la nostra Presidenza quest'anno. Il valore aggiunto dell'apposita «Dichiarazione dei Leaders sulla non proliferazione», adottata al Vertice dell'Aquila, non si esaurisce nello storico impegno dei G8 a creare le condizioni per un mondo libero dalle armi nucleari e nel forte richiamo al multilateralismo, quale cornice essenziale della collaborazione contro le armi di distruzione di massa. La Presidenza italiana ha infatti voluto sottolineare anche l'importanza della promozione di una cultura della non proliferazione e del disarmo, della formazione delle nuove generazioni e della sensibilizzazione degli scienziati che operano a stretto contatto con tecnologie e materiali potenzialmente sensibili. Uno dei caratteri distintivi dell'azione italiana nel settore della non proliferazione è la ricerca di risultati concreti. Già all'indomani della Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione del 2005, l'Italia aveva iniziato a condurre una capillare azione diplomatica per favorire un consenso su misure pratiche, non controverse, che fossero in grado di rilanciare l'agenda di disarmo e non proliferazione. Nell'ambito della Presidenza italiana del G8, ciò si è tradotto nell'impegno dei grandi a promuovere l'universalizzazione del Protocollo aggiuntivo dell'AIEA; a favorire l'entrata in vigore del Trattato contro gli esperimenti nucleari, che è ancora fermo e non ratificato dal Senato americano; a sostenere l'avvio del negoziato per un trattato che proibisca la produzione di materiale fissile per le armi atomiche. Il Trattato di non proliferazione rimane la pietra angolare del sistema di non proliferazione. Nonostante alcuni visibili limiti e le violazioni che si sono avuti a questo regime pattizio, nei 35 anni dalla sua entrata in vigore il Trattato di non proliferazione ha contribuito in modo decisivo alla pace ed alla sicurezza internazionale. È grazie al Trattato di non proliferazione se i Paesi militarmente nucleari non sono aumentati come si temeva, mentre si è ridotto negli anni il numero dei Paesi intenzionati o inclini a dotarsi dell'arma atomica. Inoltre, dobbiamo al Trattato di non proliferazione se sono stati posti in essere controlli internazionali sull'uso del materiale nucleare. L'attuale contesto internazionale ed il rinnovato impegno dei G8 ci fanno guardare con maggiore ottimismo al futuro del regime di non proliferazione, nonostante le sfide a cui tale regime viene costantemente sottoposto. Ci avviciniamo alla Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione, in programma a New York nel prossimo mese di maggio, con un capitale politico che dovrà tradursi in concreti impegni capaci di affermare l'efficacia del Trattato di non proliferazione e contestualmente rafforzare il sistema di non proliferazione. In quella sede, l'Italia agirà, di concerto con i partner dell'Unione europea, per favorire il raggiungimento del consenso tra gli Stati parte e lo sviluppo equilibrato dei tre pilastri su cui si fonda il Trattato: non proliferazione, disarmo e usi pacifici dell'energia nucleare. Lo smantellamento degli arsenali nucleari a cui ci ha richiamato il senatore Ramponi costituisce un obiettivo prioritario dell'azione dell'Italia nel campo della non proliferazione, ma insieme all'azione di Governo appare sempre più essenziale il coinvolgimento della società civile e di tutte le sedi

i partecipanti al Comitato di Oslo, tra cui vi erano ex segretari di Stato americani, come Kissinger, e il presidente Gorbaciov. ha convocato a Roma tutti gli istituti universitari delle facoltà di studi politici e strategici internazionali sul tema della non proliferazione, con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni nelle università una cultura della non proliferazione e, come si è espresso il G8, «per un mondo libero dalle armi nucleari».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il terrorismo nucleare, l'instabilità di Stati dotati ormai di armi nucleari, il mercato nero nucleare, l'espansione delle centrali nucleari e la proliferazione delle armi nucleari rappresentano minacce per tutto il mondo. Per questo, l'impegno della comunità internazionale per una loro soluzione diventa sempre più urgente, come dimostra la presa di posizione del presidente Obama nel corso del suo recente viaggio in Asia. L'approccio al dialogo e al multilateralismo di Obama sembra aver dato impulso ad un nuovo corso. Testimonianza della volontà di avviare una nuova stagione sono la Risoluzione 1887 sulla non proliferazione approvata dal Consiglio di Sicurezza, storicamente presieduto dallo stesso Presidente americano, la quale ha fatto seguito alla dichiarazione del G8 dell'Aquila per un mondo senza armi nucleari. Non possiamo non condividere la ferma condanna, da parte dei leader riuniti all'Aquila, della Corea del Nord per i test nucleari, né le preoccupazioni espresse sulla natura pacifica delle attività nucleari dell'Iran e la continua violazione dei diritti umani che si perpetra nel Paese

È auspicabile che le dichiarazioni espresse nel corso del vertice del G8 non rimangano solo tali, ma si traducano in un agire fattuale. Tuttavia, siamo consapevoli che gli Stati Uniti non possono giocare in solitaria questa sfida: essa necessita di una *partnership* globale. In particolare, decisivo appare il contributo della Federazione russa e non possiamo non plaudere all'accordo raggiunto tra i due Paesi. È necessario che l'impegno politico e le risorse dei Governi nazionali si affianchino agli sforzi della società civile, che da tempo ha preso coscienza della portata del pericolo nucleare, e si facciano più incisivi, e questo non soltanto a Natale. Tutto questo fa ben sperare, anche se, per essere realisti, la strada appare tutta in salita. Ritengo quindi, per questo, ancor più importante che anche le forze politiche italiane ribadiscano con determinazione che il solo uso possibile delle tecnologie nucleari è quello pacifico ovvero a scopi civili, che ne permetta lo sviluppo e l'utilizzo come fonte energetica, per garantire, e qui mi riferisco in particolare al nostro Paese, il superamento di quel *gap* energetico che ci vede condannati ad una condizione di non autosufficienza. Inoltre, il ricorso al nucleare, unitamente a quello alle energie rinnovabili, potrebbe concorrere a risolvere l'annoso problema del riscaldamento globale. Auspico quindi che da questa discussione, in particolare dall'approvazione dei contenuti della mozione presentata, cui il mio Gruppo ed io aderiamo, possa maturare un unanime impegno e una condivisa proposta indirizzata al Governo al fine di intensificare l'impegno dell'Italia nell'opera di disarmo

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, la trattazione di questa mozione ci permette di discutere e di riflettere su una seria e globale minaccia per la sicurezza internazionale. Dare rilievo alla questione, come facciamo qui oggi, può essere utile a tenere viva l'attenzione, e quindi l'impegno, sui principi sanciti dal Trattato di non proliferazione. Sappiamo che tra i trattati multilaterali sul controllo degli armamenti, e in particolare degli armamenti nucleari, il Trattato di non proliferazione, sottoscritto il 1° luglio 1968 ed entrato in vigore il 5 marzo 1970, è quello che ha il maggior numero di firmatari. C'è da compiacersi di come, dal 1968 ad oggi, il livello di consenso internazionale intorno al Trattato di non proliferazione sia sensibilmente e costantemente cresciuto. Elementi che contribuiscono a diminuire l'enfasi sull'opzione nucleare sono anche i Trattati START 1 e 2 sulla riduzione delle armi strategiche, la proroga a tempo indefinito del Trattato di non proliferazione e la messa a punto del Trattato di interdizione degli esperimenti nucleari, considerato indispensabile affinché gli Stati onorino seriamente l'impegno per un mondo privo delle armi nucleari. A testimonianza della validità e dell'importanza del Trattato di non proliferazione vanno citati dei casi di tentativi, fortunatamente rientrati, di proliferazione nucleare da parte di Stati non membri del Trattato: il Sud Africa Sud Africa aveva costruito una mezza dozzina di testate nucleari che ha successivamente smantellato; i tentativi di Argentina e Brasile di costruire armamenti nucleari sono stati, a quanto risulta, abbandonati. Tutti questi Paesi, infine, hanno aderito al Trattato come Stati non nucleari. Il Trattato di non proliferazione rappresenta, insomma, un pilastro fondamentale per la non proliferazione nucleare, perché fornisce la base legale non solo per la verifica internazionale È inoltre significativo che la visione sul tema sia la medesima per tutte le forze politiche; ciò sottolinea che si tratta di un obiettivo da perseguire nell'interesse nazionale e mondiale. Stati Uniti e Regno Unito si sono espressi favorevolmente; il Governo russo forse ha un atteggiamento più cauto, ma non negativo, e in Francia l'eliminazione delle armi nucleari è un obiettivo previsto dal Libro bianco della difesa. Come dicevo poc'anzi, però, l'attenzione e l'impegno devono essere tenuti vivi perché, nonostante gli importanti sforzi degli ultimi decenni, l'obiettivo della totale eliminazione degli armamenti nucleari è lungi dall'essere raggiunto. L'adesione agli impegni multilaterali nel campo del disarmo e della non proliferazione non riveste ancora un carattere universale. Si pensi che vi sono Paesi in possesso di armi nucleari che non aderiscono al Trattato e, ancor peggio, Paesi che, pur facendone parte, sviluppano attività nucleari clandestinamente. Purtroppo vige sempre la minaccia che gruppi terroristici entrino in possesso di armi di distruzione di massa, provocando una perenne preoccupazione; perciò, bisogna mettere in atto ogni sforzo possibile per impedire tale eventualità. Esistono Stati sospettati o considerati Stati nucleari ma che non si dichiarano ufficialmente tali. Fin quando esisteranno armi nucleari l'umanità correrà sempre il pericolo che vengano utilizzate o che cadano nelle mani di terroristi, minacciando la pace, la sicurezza e perfino l'esistenza umana stessa. Colleghi, personalmente sono convinto che presupposto fondamentale per la nostra riflessione sia il riconoscimento della stretta interdipendenza tra disarmo nucleare, non proliferazione nucleare e uso pacifico della tecnologia nucleare, da considerare come tre pilastri che si consolidano a vicenda. È necessaria una loro implementazione trasparente e responsabile, un progresso urgente e irreversibile su tutti i fronti, e particolare attenzione ai programmi di energia nucleare per uso civile, la cui odierna crescente espansione pone nuove potenziali sfide al regime di non proliferazione. Questo uso pacifico dell'energia nucleare dovrebbe essere sottoposto allo stretto controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Dovrebbe essere rafforzato, tramite il Trattato di non proliferazione, il potere dell'Agenzia e migliorato ulteriormente il suo sistema di vigilanza. Tutti sappiamo che la strada che condurrà all'eliminazione delle armi nucleari è lunga e si basa su specifiche condizioni politiche, la prima delle quali risiede probabilmente nell'auspicabile continuo miglioramento dei rapporti fra Stati Uniti e Russia, le due superpotenze nucleari: il loro, seppur progressivo, disarmo sarebbe un incentivo per tutti gli altri. Bisogna anelare a un vero e proprio nuovo modo di pensare. Occorre, inoltre, contribuire ad allentare le tensioni nelle aree del mondo dove è più forte il rischio che possano essere utilizzate armi o ordigni nucleari, magari a opera di gruppi terroristici (mi riferisco chiaramente al Sud-Est asiatico, India e Pakistan soprattutto, e all'area israelo-palestinese in Medio Oriente). È importante che anche l'Italia, insieme all'Europa, faccia la sua parte in questo senso. Siamo, comunque, già in grado di testimoniare che, nella nostra comunità politica tutta e in quella scientifica, vi è piena condivisione dell'importanza di questi temi e di questi obiettivi. Ribadendo, infine, che il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari è ancora una pietra angolare dei regimi di disarmo nucleare e di non proliferazione, nonché lo strumento chiave per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale, l'Italia dei Valori condivide completamente l'intenzione che il nostro Paese riaffermi continuamente il proprio sostegno al Trattato e ne esorti una sua adesione universale e la piena osservanza. Conseguentemente riteniamo opportuno che il Governo si impegni a intraprendere ogni possibile iniziativa volta a soddisfare questi obiettivi, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e attraverso contatti multilaterali e bilaterali.

importanza del 2010 sarà la Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione del nucleare. Questo documento *bipartisan* sul quale ci confrontiamo prende atto, secondo me, di una fondamentale realtà: il primo periodo

nucleare esercitata in quegli stessi anni da Israele, è di fatto cominciata con la doppia tornata di esperimenti condotta a Nuova Delhi e in Pakistan nel 1998.

Sapevamo che gli americani e i sovietici, ed in minore misura i francesi, i cinesi e i britannici, possedevano ingenti quantitativi di armi di eccezionale capacità distruttiva,

hanno poca affidabilità e mostrano una razionalità strategica molto dubbia. Una delle ragioni che secondo noi hanno obbligato gli Stati Uniti, i loro alleati e tutti noi ad occuparci dell'Afghanistan

come moneta di scambio; è un altro aspetto negativo di ciò che si va profilando in questo decennio,

confermare i tradizionali orientamenti della politica estera italiana in campo nucleare: dobbiamo avere la piena consapevolezza dell'esigenza di confermare la strada che stiamo perseguendo. Il nostro Paese, a mio avviso, ha messo in

Siamo ovviamente consapevoli che il disarmo completo e definitivo è destinato a rimanere un obiettivo di lungo respiro: però dobbiamo essere mossi dall'idea che la direzione che stiamo percorrendo è quella giusta. Si tratta altresì di enunciare dei punti di riferimento che saranno utili anche per tracciare il percorso politico da seguire nelle eventuali trattative con l'Iran e con tutti i Paesi che lo seguiranno

battersi per un mondo libero dagli ordigni atomici significa sicuramente non solo rafforzare gli attuali regimi di non proliferazione, ma riguarda anche la controproliferazione nucleare, nell'adottare un atteggiamento molto fermo nei confronti di chi vuole continuamente fare ricerca su questo settore. Riteniamo che questo debba essere uno strumento per rivendicare

quindi che lavorare sui giovani sia la cosa migliore rispetto alle reprimende che facciamo noi, se volete anche in Parlamento - lo dico Sono i giovani che devono imparare e capire profondamente il segnale che vogliamo dare. Condivido l'importanza di confermare l'impegno del nostro Paese Abbiamo visto in particolare con gli esperimenti condotti dalla Repubblica popolare cinese che ci sono stati grossi problemi.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mozione sulla non proliferazione di armi nucleari ha dato modo di affrontare un'altra volta, con rinnovato rigore, una problematica che ha costantemente coinvolto l'opinione pubblica mondiale dal termine del secondo conflitto mondiale fino ad oggi. L'ha coinvolta suscitando in essa percezioni diverse: dall'iniziale sentimento di terrore per una minaccia immanente ed incombente di impiego degli ordigni nucleari - era il periodo della deterrenza nucleare e della guerra fredda alla speranza di un accantonamento delle armi di distruzione di massa, dalla successiva illusione di poter bloccare la diffusione di quelle armi, limitando la disponibilità a pochi Paesi, fino alla sconfortante presa d'atto del diffondersi delle capacità tecnologiche sufficienti per realizzare nuovi ordigni distruttivi. In particolare, gli anni che vanno dalla fine della guerra fredda ai nostri giorni hanno visto non solo nascere una nuova generazione di conflitti, i conflitti asimmetrici, che hanno comportato la necessità di rivedere i vecchi parametri della guerra convenzionale, ma anche ridursi la speranza di accantonare gli arsenali nucleari dei Paesi che ne dispongono di fronte alla determinazione di altri Paesi che, non disponendone, davano corso all'acquisizione di assetti e procedimenti per lo sviluppo di tecnologie nucleari, talvolta proprio per uso militare. Certamente, la consapevolezza della pericolosità di una siffatta situazione suscettibile di gravi rischi per la sicurezza generale ha indotto i Paesi di maggior peso politico e strategico a ricercare accordi che coinvolgessero anche i Paesi non detentori della tecnologia militare. Il Trattato di non proliferazione del 1970 è stato il primo passo per porre sotto controllo il settore nucleare, ma anche il Trattato START 1, in vigore dal 1994, aveva lo stesso scopo, così come lo START 2, ratificato nel 1996, ed ancora il Trattato per la completa messa al bando dei*test* nucleari dello stesso 1996, ma accolto solo da poche Nazioni e, infine, il Trattato di Mosca del 2002. In sostanza, 40 anni di iniziative e di tentativi spesso avviati e sviluppati in un clima di diffidenza ideologica che purtroppo non sono pervenuti alla neutralizzazione della minaccia nucleare; minaccia che, anche se non è più incombente come durante la contrapposizione dei blocchi ideologici e politici, rimane pur sempre immanente, se è vero, com'è vero, che l'accordo START tra Stati Uniti e Russia scade nel corrente mese di dicembre e dovrà essere rinegoziato. E ancora, se è vero, com'è vero, che il numero dei Paesi detentori di ordigni nucleari è sensibilmente aumentato, inglobando Nazioni appartenenti ad aree di crisi continua, come il Vicino, il Medio e l'Estremo Oriente, con tutte le rischiose conseguenze che ciò comporta: penso naturalmente al Pakistan e all'India, penso alla Corea del Nord, a Israele e, chissà, nel futuro forse dobbiamo pensare all'Iran e alla Siria. Ma non è solo la consapevolezza che gli armamenti nucleari sono ormai nella effettività disponibilità di numerosi Paesi, talvolta non perfettamente integrati nel sistema dei rapporti internazionali o addirittura portatori di politiche aggressive, a rendere concreto il pericolo degli armamenti nucleari. Infatti, il rinnovato interesse per l'energia nucleare civile da parte di un crescente numero di Nazioni decise ad avviare programmi di sviluppo di tale energia alza fortemente i rischi di deriva della ricerca verso obiettivi e finalità di carattere militare. In definitiva, c'è la necessità di un ulteriore forte impegno per mantenere nei limiti del consentito l'utilizzazione dell'energia nucleare e per ridurre il pericolo degli ordigni nucleari. Allora dobbiamo accogliere con grande favore le iniziative delle Nazioni Unite che, con una specifica risoluzione, hanno invitato tutti gli Stati a sottoscrivere e a rispettare il Trattato di non proliferazione. Dobbiamo accogliere con grande favore, altresì, la determinata azione del presidente Obama che sin dalla sua elezione ha fatto della battaglia alla non proliferazione nucleare un suo obiettivo primario. In tale contesto ben venga, inoltre, il continuo stimolo dell'Unione europea che solo qualche mese fa ha elaborato e diramato a tutti i Paesi una nuova efficace direttiva per la non proliferazione. Ben venga, ancora, il sostegno all'Agenzia internazionale per l'energia atomica che svolge, attraverso le attività di controllo disciplinate dal Trattato di non proliferazione, un ruolo fondamentale nell'impedire deviazioni dai programmi di utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici. Ben venga infine la mozione di cui oggi discutiamo, che ha come prima firma quella del senatore Ramponi e che è stata presentata congiuntamente da tutti i Gruppi del Senato, per impegnare il Governo ad un'azione incisiva in campo internazionale e dipolomatico per ridurre o accantonare gli armamenti nucleari, salvaguardando anche spazi, come quello extra-atmosferico, che sono ancora immuni dalla presenza di ordigni nucleari. una mozione che è completamente in armonia con le numerose iniziative di moderazione che hanno sempre caratterizzato la politica del nostro Paese nel campo della ricerca della pace e del rispetto dei diritti umani. Basti ricordare al riguardo che l'Italia e' stata tra le primissime Nazioni a bandire l'impiego e la costruzione delle mine antiuomo, che tante vittime mietono purtroppo ancora oggi tra la popolazione civile. Basti ricordare altresì che proprio il Senato, all'inizio della corrente legislatura, ha approvato uguali misure nei confronti dell'altra piaga rappresentata dalle *cluster bombs* o bombe a grappolo. Sono decisioni di civiltà che credo debbano inorgoglirci. Allo stesso modo, dobbiamo manifestare soddisfazione per la moratoria della pena di morte che l'Italia ha promosso nell'ambito delle Nazioni Unite qualche anno fa o per la salvaguardia dei diritti umani, che vede il nostro Paese sempre in prima fila. Per questi motivi, il Partito Democratico esprime il suo convinto sostegno alla mozione sulla non proliferazione degli armamenti nucleari, e naturalmente annuncia mio tramite il voto favorevole, augurandosi che il Governo, forte anche del generale consenso che otterrà il documento, riesca ad operare efficacemente, come tutti auspichiamo, in campo internazionale e diplomatico per l'eliminazione del pericolo rappresentato dall'incredibile numero di ordigni nucleari ancora presenti nel mondo; lo voglio ricordare, è ben superiore a quello sufficiente per compromettere la stessa esistenza della nostra civiltà.

Presidente, a nome del nostro Gruppo dichiaro il voto favorevole, ma mi sembra pleonastico, dal momento che questa mozione è originata proprio in seno al PdL. Le ragioni per le quali voteremo in senso favorevole, o meglio, per le quali abbiamo presentato questa mozione, sono già state da me in precedenza indicate e poi via via sostenute da tutti i colleghi che hanno preso la parola, confermando una sostanziale convergenza sul documento. Farò soltanto riferimento a un paio di punti

Il secondo punto che voglio illustrare è di carattere squisitamente politico. Tutto il mondo è interessato

Ebbene, questo impegno nei confronti dell'Iran da parte dell'Unione europea, del gruppo dei Cinque, degli Stati Uniti e della Russia può trovare una *audience* ed avere un sostegno in in termini di coscienza pulita nel caso in cui venga sviluppata una autentica azione di riduzione degli ordigni, una autentica conferma di non proliferazione,

non avere l'ordigno nucleare. Una delle ragioni per cui deve essere molto serio questo impegno - come avete tutti auspicato - a dare vita ad iniziative di riduzione è proprio il fatto che, se vogliamo avere la coscienza pulita nei confronti dell'Iran, dobbiamo, noi per primi, dare l'esempio

tale mozione. Essa nasce da un convegno che io stesso ho organizzato, nell'ambito del quale il concetto ispiratore di questa mozione è stato sottoposto non solo al giudizio giudizio - comunque estremamente opportuno - di tutti i Capigruppo del Senato (un giudizio politico che li ha visti convergenti

Mi rimangono pochi minuti per fare una considerazione che è *a latere*, ma che ritengo ugualmente importante. Tutti avete detto che una delle valenze politiche è la convergenza - il Senato compatto - su una indicazione di grandissima importanza che sollecita il nostro Governo ad essere protagonista - nella misura in cui il peso politico ed economico della nostra Nazione si manifesta nel mondo - su questa iniziativa, che è è uno degli argomenti che assilla la società mondiale. Ebbene, questa convergenza deve essere esemplare. La mozione non nasce a seguito dell'ultimo fatto deprecabile. Nasce prima. Nasce dalla mia personale convinzione che vi è abbondante spazio per trovare luoghi, punti nei quali entrambi gli schieramenti, maggioranza e - non la voglio chiamare opposizione - minoranza, possano svolgere una funzione positiva, di stimolo per il Governo, di approvazione di emendamenti e di leggi, uniti, anziché cercare disperatamente elementi di contrasto, quel no continuo che diventa addirittura quasi ridicolo. La mozione dimostra questo. Invito tutti a fare una riflessione. Il fatto che in Senato si sia trovata questa convergenza è negativo per qualcuna delle componenti, maggioranza o minoranza, agli occhi della nostra popolazione? Direi proprio di no. Se andassimo ad interrogarli con Piepoli, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani direbbero che sono soddisfatti perché abbiamo lavorato bene assieme a favore della nostra società e della pace mondiale.

dibattito e alla continua negazione di ogni iniziativa, da una parte e dall'altra. Voglio dire: per trovare un equilibrio nei rapporti politici italiani non credo sia necessario

Mi riferisco ad una frode che non è stata consumata dal mariuolo di turno, ma da un'importante banca che è coinvolta nel progetto Brontos. Secondo un'indagine del pubblico ministero di Milano, Afredo Robledo, UniCredit avrebbe messo in atto una sofisticata operazione di pronti contro termine mediante un *software* della Barclays Bank, concretizzando reati di elusione, evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato per un controvalore di 250 milioni di euro, ossia 500 miliardi

alle domande e, anzi, rappresentando una situazione idilliaca circa i rapporti con i cittadini e le piccole e medie imprese, persino offensiva dell'ordinaria intelligenza. Questi signori banchieri, direttamente responsabili della grave crisi economica